il decreto-legge in esame contiene una serie di modifiche che concernono il codice penale e il codice di procedura penale, oltre ad una serie di norme strutturali di corredo che comunque attengono a problematiche di ordine pubblico e sicurezza. In particolare, all'articolo 1 viene sostanzialmente reintrodotta l'aggravante di cui al numero 5) dell'articolo 576 del codice penale in cui vi era il riferimento ai reati contro la moralità pubblica che poi sono stati abrogati.

persona offesa, ma che può essere anche sanzionato d'ufficio nei casi aggravati, cioè se viene condotto nei confronti di minori

Nel caso prosegua in questo suo comportamento, evidentemente il reato sarà perseguibile d'ufficio. Vi sono poi una serie di modifiche del codice di procedura penale - in particolare mi riferisco al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale - che riguardano

aggiunti tutti i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quarter*, con un significativo ampliamento con riferimento alle associazioni a delinquere semplici, alle associazioni a delinquere contemplate contemplate dalla legislazione speciale, alla tratta e riduzione in schiavitù delle persone, al sequestro di persone e a reati di terrorismo. Vengono altresì aggiunti

del codice di procedura penale vengono altresì estese ai delitti di violenza sessuale, violenza sessuale nei confronti di minori e violenza sessuale di gruppo, purché non ricorrano le attenuanti specificamente indicate per questi reati.

Sappiamo che la regola generale prevede l'arresto in flagranza per reati che prevedano una sanzione punitiva di un minimo di cinque anni e di un massimo di 20 anni o dell'ergastolo.

l'introduzione dell'incidente probatorio fuori dalla regola generale con riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572) e di atti persecutori relative modifiche riguardo all'articolo 398 del codice di procedura penale, che prevede il provvedimento su richiesta dell'incidente probatorio. Viene prevista poi la possibilità di esame delle vittime minori o maggiorenni inferme di mente attraverso il vetro, così come indicato dall'articolo 498 del codice di procedura penale.

dall'elenco esistente nel comma 1 vengono eliminati l'articolo 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (violenza sessuale aggravata) e 609-*quater* (atti sessuali su minori). Viene mantenuto l'impianto del precedente comma 1 nel comma 1-*bis* e nel comma 1-*ter* viene eliminato l'articolo 609-*quater*

commesse nell'ambito associativo per le quali, in caso di collaborazione, è possibile accedere a determinati benefici penitenziari. Ebbene, da tale elencazione vengono eliminati i reati a cui ho appena accennato. Infine, viene aggiunto il comma 1-*quater*, che prevede che i benefìci di cui al comma 1 concessi, per i reati di violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, violenza sessuale su minori e violenza sessuale di gruppo, solo dopo un procedimento di osservazione della personalità, svolto da un collegio specificatamente indicato, della durata di almeno un anno. Con l'articolo 4 si modifica il Testo unico in materia di spese di giustizia con l'ammissione al gratuito patrocinio delle vittime di violenza sessuale (609-*bis*), violenza sessuale su minori (609-*quater)* e violenza sessuale di gruppo (609-*octies*), anche in deroga al livello di reddito

per 100 milioni di euro, alle necessità urgenti delle forze dell'ordine per quanto attiene all'attività di controllo del territorio. infine ripristinato con la somma di 3 milioni di euro il progetto per il fondo di assistenza per le vittime della violenza sessuale. Vi è poi l'interpretazione autentica per quanto riguarda l'elenco dei proventi dei beni sequestrati e confiscati, dai quali vengono esclusi i proventi dei complessi aziendali. prevista l'utilizzazione dei servizi di videosorveglianza da parte dei Comuni in luoghi pubblici e aperti al pubblico con conservazione dei dati per sette giorni, salvo eventuali esigenze di conservazione ulteriore (naturalmente su richiesta dell'autorità giudiziaria o di altra autorità). l'immissione in servizio permanente presso l'Arma dei carabinieri di ufficiali attualmente in servizio in ferma breve, cioè per la durata di tre anni, attraverso una relativa procedura concorsuale con la previsione che, nelle more dell'espletamento del concorso, l'Arma dei carabinieri possa continuare ad utilizzare anche dopo il termine indicato gli ufficiali che si trovano in questa situazione. Con l'articolo 10 viene aumentata la durata del cosiddetto ordine di protezione, contenuto nell'articolo 342-*ter* del codice civile, da sei mesi a un anno. dell'ordine di allontanamento dalla residenza familiare, dell'ordine di cessazione di azioni nei confronti di coniugi o di prole e dell'intervento dei servizi sociali. Viene poi realizzato un obbligo di informazione sui centri antiviolenza esistenti da parte di forze dell'ordine, presidi sanitari e altre istituzioni pubbliche con le quali entrano in contatto le vittime di reati di *stalking*, di violenza sessuale e di abuso in generale. Su richiesta della stessa vittima si realizza da parte di questi organismi il contatto diretto con questi centri antiviolenza istituiti. Con l'articolo 12 viene istituito un numero verde di prima assistenza, di consulenza giuridica e di sostegno psicologico presso il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attivo 24 con un rapporto diretto di comunicazione alle forze dell'ordine. Nella sostanza delle cose, si consente alla vittima di evitare un'esposizione diretta attraverso una denuncia

denuncia della comunicazione telefonica intercorsa con la vittima, le forze dell'ordine potranno intervenire per verificare quanto avviene. Con l'articolo 12-*bis*, vengono escluse per il personale delle forze di polizia e delle Forze armate le norme in tema di assicurazione sul lavoro, cioè la normativa di carattere generale al riguardo, in relazione alla specificità alla specificità e alla particolarità dell'attività svolta da questo tipo di personale della pubblica amministrazione, rinviando agli ordinamenti esistenti (quindi non vi è un vuoto normativo) e in attesa del riordino complessivo della materia. Con l'articolo 12-*ter* vengono poi affrontate alcune problematiche relative ai dati della comunicazione e alla loro conservazione e messa a disposizione. Evidentemente, parliamo anche con riferimento allo stesso articolo 612-*bis*, che viene introdotto con l'indicazione di alcune scadenze. Infine, l'articolo 13 prevede la delega al Ministro dell'economia e delle

Signora Presidente, ancora una volta il Governo ci impone misure di inasprimento di pena in un contesto in cui in Italia ormai lo Stato di diritto non esiste più. Quotidianamente siamo confrontati con la patente illegalità costituzionale per cui i diritti civili e politici degli italiani - indipendentemente dal contesto o dall'ambito in cui essi si trovino - non sono non sono godibili, perché le istituzioni stesse sono le prime ad agire contro le proprie leggi. Sebbene alla Camera dei deputati abbiamo visto un sussulto di ragionevolezza che ha fatto cancellare almeno due delle pessime misure che rientravano in quella versione del decreto (cioè le ronde e la permanenza fino a sei mesi all'interno dei CIE), la delegazione Radicale del Gruppo del Partito Democratico qui al Senato ritiene che anche questa versione, depurata da queste due pessime misure, sia da respingere totalmente, abbiamo proposto due pregiudiziali di costituzionalità. Riteniamo infatti che estendere, come previsto all'articolo 2, tutta una serie

La modifica in discussione comporta la compressione delle libertà personali nella modalità più estrema (cioè la custodia cautelare in carcere), per una molteplicità di condotte assai eterogenee, sottraendo del tutto al giudice e il relatore era un magistrato, una volta - la valutazione di adeguatezza della misura. Un simile meccanismo è peraltro funzionale al cosiddetto fenomeno di anticipazione della pena, che diviene paradossalmente effettiva (conoscendo i tempi della giustizia italiana, criminale abituale sanzionato quotidianamente dalla Corte di Strasburgo dei diritti umani), proprio perché irrogata senza processo, proiettando un'immagine dimidiata del diritto al processo,

Non si è in presenza di una situazione di fatto di tale natura atteso che il provvedimento in esame viene motivato, nel preambolo, essenzialmente sulla base della crescita dei casi di violenza sessuale, mentre dai dati che sono stati comunicati dal Viminale proprio il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto-legge, si ricava come nel corso del 2008 vi è stata una non indifferente diminuzione di questi episodi criminosi rispetto all'anno precedente (meno 8,4 per cento). Ciò ovviamente non significa che da parte nostra non ci sia grande

le disposizioni che caratterizzano questo decreto-legge (cioè quelle penali e processuali in materia di violenza sessuale) sono state estrapolate dal disegno di legge n. 733, già approvato dal Senato e attualmente in discussione alla Camera dei deputati, siamo nella situazione paradossale per cui il Parlamento rischia di approvare una legge dai medesimi contenuti del decreto in esame prima di affrontare la legge di conversione di quest'ultimo, ovvero, viene costretto ad ad emendarne il testo, costringendo inevitabilmente il disegno di legge ad una seconda lettura al Senato, per espungere le disposizioni già anticipate dal Governo. Siamo davvero di fronte a un corto circuito legislativo che getta più di qualche ombra sull'effettiva rispondenza del decreto in esame ai requisiti posti dalla Costituzione per la sua adozione e fornisce la misura dell'attuale crisi dei rapporti tra Esecutivo e Parlamento in ordine all'esercizio della potestà legislativa, così come scolpiti nella legge fondamentale.

consiste in maggiori pene, ergastoli, nuove fattispecie di reati, doppi binari processuali, smantellamento della legge Gozzini e dei benefici penitenziari, cattura obbligatoria e carcere in violazione della presunzione di innocenza e abuso dell'incidente probatorio.

i due presupposti richiesti per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, cioè i gravi indizi di colpevolezza e l'assenza di elementi dai quali possa risultare l'insussistenza di esigenze cautelari. tali norme sono frutto di un bilanciamento intelligente fra le esigenze di tutela della libertà personale - che non vengono assolutamente intaccate - e l'esigenza di tutela della collettività. Esistono poi, all'interno di questo provvedimento, norme particolarmente importanti, frutto di emendamenti proposti dal nostro Gruppo. Mi riferisco, per esempio, alla possibilità di utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di conservare le immagini determinate da questi impianti per almeno sette giorni. Oggi la disciplina è lasciata ad un provvedimento amministrativo, ad una deliberazione del Garante, che ha fissato discrezionalmente un termine eccessivamente breve: per non più di ventiquattr'ore possono essere conservate queste immagini.

la consumazione dei reati in materia di violenza sessuale è certamente - questo è un dato di comune esperienza - favorita dalla presenza dei clandestini e dalla insufficienza dei controlli sul nostro territorio. Quindi, dobbiamo riflettere su quella parte che purtroppo non troviamo più all'interno di questo provvedimento, in parte cassata - possiamo usare questo termine - dalla Camera dei deputati. alla parte relativa ai termini di trattenimento dei clandestini all'interno dei centri di identificazione e di espulsione. Su questo provvedimento abbiamo presentato un ordine del giorno, che vuole impegnare il Governo a dare attuazione alla direttiva comunitaria 2008/115/CE sui rimpatri, una direttiva comunitaria che sui termini di trattenimento dei clandestini all'interno dei centri di identificazione e di espulsione è molto più rigorosa molto più rigorosa della norma che era contenuta nel decreto-legge e che, grazie all'emendamento Franceschini (ovviamente il termine "grazie" è eufemistico), è stata eliminata da questo provvedimento. La direttiva europea - spesso in Aula ci si riempie la bocca di europeismo, ma a senso unico e non si comprende che sovente le normative comunitarie debbono essere applicate ed attuate indipendentemente dal convincimento delle opinioni personali personali - prevede che il tempo di trattenimento dei clandestini all'interno dei centri sia non superiore a sei mesi: ed è esattamente quello che prevedeva la norma contenuta nel decreto-legge,

Ma la stessa direttiva 2008/115/CE prevede che questo periodo dei sei mesi possa essere superato per ulteriori 12. Arriviamo così a 18 mesi, nel caso in cui -leggo testualmente la direttiva - «nonostante siano stati compiuti tutti gli sforzi che sia lecito aspettarsi, l'operazione di allontanamento dei clandestini rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del clandestino oppure dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi di origine». Quindi, la direttiva ci dice che se il clandestino non collabora ai fini della sua identificazione o se il Paese d'origine del clandestino non fornisce documenti, il clandestino può essere trattenuto fino a 18 mesi. Dunque, 6 più 12: 18 mesi Ma questa direttiva aggiunge che tale trattenimento deve avvenire di norma in centri di permanenza temporanea, ma possa avvenire anche in istituti penitenziari, purché i clandestini siano tenuti separati dai detenuti ordinari;

inequivocabilmente un numero eccezionalmente elevato di clandestini da rimpatriare): cioè, in tali situazioni il requisito del trattenimento separato dei clandestini in carcere rispetto ai detenuti ordinari può venire meno.

noi ora chiediamo che la direttiva venga attuata integralmente, come deve essere, come ogni provvedimento comunitario che viene attuato in quest'Aula, anche per evitare che accada quanto potrebbe accadere fra pochi giorni, grazie all'emendamento Franceschini, e cioè quasi 1.300 clandestini siano rilasciati dai centri iniziando a vagare sul nostro territorio, senza un'identità, senza sapere che cosa fanno e spesso diventando manodopera della criminalità più o meno organizzata, e magari diventando anche autori di reati a sfondo sessuale (perché questo ci dicono le statistiche giudiziarie). Ecco, per tutti questi motivi motivi voteremo a favore di tale provvedimento, ma chiediamo anche un serio impegno per evitare che la questione del trattenimento dei clandestini nei centri di identificazione e l'efficacia delle procedure di espulsione non vengano poste nel nulla.

Sono problemi sui quali la convergenza andrebbe sempre cercata, voglio aggiungere, a tutti costi, anche quando non dovesse esserci all'inizio. Le misure previste sono diventate sempre più necessarie, lo sappiamo, e ci siamo sempre adoperati perché si potesse arrivare a delle leggi efficaci nel tempo più breve possibile. I casi di violenza sono davvero troppi. Sono troppi i casi di stupro da parte di sconosciuti; spesso si tratta di stupri di gruppo, come quelli recenti, su donne giovanissime accompagnate dai loro *partner*. Sono troppi anche i casi di violenze esercitate in famiglia (quasi l'80 per cento); non dobbiamo mai dimenticare questo dato: magari questi casi non arrivano alla cronaca perché sono vissuti nel silenzio, nel chiuso delle mura domestiche. Per quanto riguarda lo *stalking*, le vittime sono oltre 2.000.000. È importante che si arrivi, come il provvedimento in discussione prevede, al riconoscimento della fattispecie di reato così da garantire il diritto delle persone a vivere liberamente la propria vita e le proprie scelte, senza arrivare a rischiarla o a vivere nell'angoscia.

(si può fare sempre di più) e credo che di più si debba e si possa fare tutti, nell'investimento di risorse che sono davvero scarse, come copertura di questo provvedimento, e nella prevenzione. Vogliamo insistere su questo punto: la prevenzione è la parola chiave in questa materia e per questi problemi. Prevenzione vuol dire formazione, vuol dire educazione al rispetto reciproco fra uomini e donne. Quando si parla di violenza sessuale si pensa che sia una questione di cui debbano occuparsi le donne. Certo, le donne sono il più delle volte le vittime, ma il problema vero riguarda le modalità di convivenza fra uomini e donne, la relazione

«La violenza di genere e tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e perciò devono essere eliminate». E ancora, nella piattaforma di Pechino del 1995: «La violenza contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di eguaglianza, sviluppo e pace. La violenza contro le donne viola, indebolisce o vanifica il godimento da parte delle donne dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali». Quindi, noi oggi stiamo facendo qualcosa di davvero importante a salvaguardia della tutela della dignità della donna e della dignità della persona. che tutti e tutte abbiano in mente il dolore, lo sconcerto e lo smarrimento di quelle donne che hanno subito violenza e che non sanno se riusciranno mai a ripartire e a riprendere in mano la loro vita. Vogliamo che non siano mai sole, che possano sempre disporre di un luogo in cui cercare e trovare solidarietà, assistenza, sostegno per ritrovare se stesse e riacquistare dignità,

Signora Presidente, intervengo per chiedere alla Presidenza di voler valutare la possibilità di far conoscere all'Aula il contenuto della lettera che il Presidente della Repubblica

Signora Presidente, il nostro Gruppo, così come è avvenuto alla Camera, ha ritenuto di

che la norma qualificante di questo provvedimento, ossia gli atti persecutori, è materia di esame del Parlamento,

decisione volta ad introdurre nel nostro codice un reato che va a colmare quel cono d'ombra riguardante determinati comportamenti non diversamente aggredibili. Ciò che dispiace è il fatto che un decreto‑legge, per il quale è previsto un termine di conversione di 60 giorni, sia assegnato a quest'Aula e a questo ramo del Parlamento cinque giorni prima della imposta imposta conversione (perché decade se non si approva entro il 25 aprile). Ed è un peccato, perché questo ramo del Parlamento è stato privato della possibilità di interloquire, di intervenire con delle modifiche che sarebbero state opportune. Non possiamo esercitare questo potere per cui o insistiamo

sarebbe stato estremamente importante e rilevante, perché il testo che ci è stato consegnato dalla Camera è un testo

di un ragazzino o di una ragazzina infradecenne la pena vada da sette a quattordici anni. Si prevede cioè la misura cautelare come misura principale. Non capisco perché, intervenendo sull'articolo 380, ossia sull'arresto obbligatorio in flagranza,

perché i tempi non ce lo consentono. Così come la previsione

un gravissimo errore in quanto, proprio per la tipicità dei fatti persecutori, rendendo il reato perseguibile su querela, che si può presentare entro sei mesi, si espone ancor

qualora la persona venga arrestata, subisca un periodo di carcerazione preventiva e poi la parte offesa ritiri la querela, rendendo improcedibile il reato.

Ma possiamo noi dimenticare che la Corte costituzionale ha eliminato gli articoli da 157 a 164 del Testo unico di pubblica sicurezza, che prevedevano l'ammonimento, in quanto ha ritenuto che ai sensi dell'articolo 13 della nostra Carta costituzionale simili provvedimenti debbano avere natura giurisdizionale e non amministrativa? Noi, invece, abbiamo rispolverato un istituto che contiene un atto amministrativo, ossia l'ammonimento, assegnando però allo stesso una ricaduta sul piano processuale; il reato, infatti, diventa procedibile d'ufficio qualora la persona querelata sia stata in precedenza ammonita. Un atto amministrativo, quindi, diventa condizione di procedibilità d'ufficio. Non solo, si introduce anche l'aggravante per colui che commette atti persecutori qualora sia stato attinto da un provvedimento di ammonizione. ci si dimentica di specificare se l'ammonizione debba riguardare un atto persecutorio nei confronti della medesima persona.

dobbiamo stigmatizzare è l'espropriazione delle prerogative del Parlamento per cui disegni di legge d'iniziativa parlamentare vengono fatti propri dal Governo, sotto forma di decreto,

come ci sia poco rispetto per il Parlamento, per il nostro lavoro e per il contributo che ognuno di noi può offrire a provvedimenti che si presentano certamente come importanti.

Questo un po' mi dispiace perché alla fine l'articolo 46 tratta un argomento molto serio, molto attuale e molto sentito da tutti i cittadini: parla di sicurezza partecipata,

come bisogno primario di una vita democratica. Il tema della sicurezza è sentito, credo, fortissimamente in questo periodo perché

fanno diventare quanto mai attuale e drammatico il tema della sicurezza. Allora, cosa fare? Credo che il nostro Ministro dell'interno qualcosa di positivo l'abbia fatto in questi ultimi dodici mesi. I risultati sono evidenti, forti e chiari. Si parla sempre più spesso di grandi risultati da parte delle forze dell'ordine e in questo colgo l'occasione per complimentarmi con loro. Anche gli stanziamenti nei confronti delle Forze dell'ordine,

parlava tanto, ma concretizzava poco. Finalmente in questi ultimi dodici mesi nei confronti delle forze dell'ordine gli investimenti strutturali sono aumentati. Ma questo non basta assolutamente. Ecco allora che i sindaci, che in questo ultimo periodo hanno nuove e molto più importanti competenze in quanto a controllo del territorio, si erano inventati il controllo del territorio con la sicurezza partecipata con i cittadini. Non vi è nulla di strano, tutto è solo ed esclusivamente molto positivo. Si tratta semplicemente di una sorveglianza attiva con dei volontari che alla sera vanno in giro per il territorio controllati dai sindaci,

Non sto facendo retorica perché sono dati del Viminale: centinaia e centinaia di sindaci hanno adottato e stanno controllando il territorio con questo sistema.

prefetto, per il territorio a vedere che non ci sia il reato di abigeato, il furto di bestiame. Sono ben 111 anni che le ronde stanno funzionando in Sardegna. Sardegna. Se da 111 anni in Sardegna questo sistema partecipato di controllo del territorio sta funzionando, mi risulta difficile capire il motivo per cui non possiamo farlo in tutta Italia e non possiamo rendere legittima una forma di volontariato che già si sta rendendo utile e che può solo dare una mano per combattere la criminalità dilagante. Purtroppo la demagogia di sinistra,

questi onorevoli e questi senatori dovranno rispondere alle loro coscienze e ai loro cittadini elettori. Signora Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo dare atto dello sforzo comune che è stato fatto per portare rapidamente all'approvazione definitiva alcune disposizioni molto importanti, che da tempo erano attese: mi riferisco alle norme che introducono la nuova fattispecie delittuosa del reato di atti persecutori. Questo tema da tempo, anche nel nostro Paese, generava e genera allarme e preoccupazione. L'esperienza di ciascuno di noi e la cronaca più recente ci dicono da tempo che molte persone sono vittime di comportamenti molesti altrui che, anche quando non sfociano in gesti gravemente lesivi, condizionano però pesantemente la vita delle vittime, procurano loro stati di preoccupazione, angoscia e paura, che le vecchie norme sulle molestie e la violenza privata non erano idonee a prevenire. Da una parte, infatti, la previsione legislativa sulle molestie presuppone una condotta di modestissima gravità, prevede una pena mite e non consente di adottare misure cautelari; dall'altra parte la previsione normativa riferita alla violenza privata richiede, per la sussistenza dell'elemento materiale, fatti di violenza o minaccia che spesso mancano nella condotta di chi piuttosto pone in essere atti di disturbo, di condizionamento, magari atti non violenti ma che spesso progrediscono fino a diventare gravissimi. La realtà sociale di cui riferiscono le cronache parla di persone che decidono di non avere o di non avere più rapporti con altre, perché si tratta di coniugi che si sono separati, o di una relazione sentimentale interrotta interrotta o mai iniziata perché solo uno dei due la desidera. Queste persone spesso si trovano intrappolate in una rete di comportamenti molesti, con cui l'altro vorrebbe convincerle a mutare atteggiamento o messi in atto per mero spirito di vendetta: telefonate anonime o mute, spesso ripetute più volte al giorno; appostamenti sotto l'abitazione o presso il luogo di lavoro; messaggi al cellulare; lettere e piccoli danneggiamenti. Condotte che in sè contengono un'offensività modesta ma che, se ripetute ossessivamente nel tempo, costringono la vittima a modificare le proprie abitudini, a vivere con il sospetto e a temere un intensificarsi delle aggressioni. se poste in essere da individui che non mantengono appieno il contatto con la realtà e il controllo dei propri sentimenti, queste sono condotte che spesso conducono a fatti ben più gravi, a delitti o tentati delitti di omicidio o lesioni. Le vittime più numerose di queste condotte, anche se non sono le uniche, sono naturalmente le donne, che sono spesso moralmente più forti e coraggiose nel porre fine a relazioni o nel rifiutare contatti, ma anche più vulnerabili rispetto ad una violenza subdola o aggressiva. Apprezziamo pertanto che la maggioranza abbia deciso di farsi carico di questo problema e, unificando progetti e proposte legislative di diversa provenienza, abbia permesso di portare a compimento una riforma importante e significativa: anch'io avevo presentato un disegno di legge in proposito nella scorsa legislatura. Apprezziamo anche il fatto che, raccogliendo anche in questo caso proposte e suggerimenti di varia origine mi riferisco in particolare alla proposta formalizzata dal governo Prodi nel 2007 con il disegno di legge sulla violenza nelle relazioni familiari - le misure previste dal decreto‑legge n. 11 non si limitano ad introdurre un nuovo reato, ma aggiungono norme preventive riguardanti comportamenti precedenti alla denuncia da parte della persona offesa, introducono disposizioni cautelari con misure e divieti appositi, disposizioni processuali, interventi sociali da parte della collettività, misure a sostegno delle vittime. Rilevo in particolare l'utilità, se ben applicata, di una misura quale quella dell'ammonimento, disposta dal questore quando i fatti non sono ancora tanto gravi da configurare il reato. Era prevista anche nella mia proposta di legge, perché era finalizzata proprio ad evitare sia l'apertura di procedimenti penali nei casi che possono risolversi invece bonariamente, sia che certe condotte degenerino in fatti più gravi. Casi che spesso l'intervento dei privati non è sufficiente ad arginare. L'ammonimento, oltre a valere in sé come atto dall'effetto dissuasivo, ha giustamente l'ulteriore effetto di aggravare il fatto persecutorio commesso successivamente, rendendolo procedibile anche d'ufficio. Certo, il testo dovrà essere migliorato, soprattutto per far sì che nelle aule di giustizia non sorgano né problemi interpretativi né ostacoli all'applicazione concreta della nuova normativa.

dovremmo rammaricarci che il confronto politico su una questione tanto seria e impellente quale l'emergenza sicurezza cada proprio nel periodo in cui incalzanti e fuorvianti premono le necessità della propaganda di partito. Con l'approssimarsi della scadenza elettorale, infatti, subisce un ulteriore ridimensionamento il già non eccelso grado di onestà intellettuale dimostrato da quanti si sono scagliati contro due provvedimenti di palese buon senso, che hanno invece piena legittimità e ampia condivisione da parte dell'opinione pubblica. Mi riferisco, come hanno già fatto altri colleghi, alle misure finalizzate a riconoscere e regolarizzare il volontariato civico in materia di sicurezza e al provvedimento che consente l'effettiva espulsione degli immigrati clandestini. Specialmente intorno al primo punto abbiamo assistito ad un dibattito del tutto surreale, in cui si sono sprecate accuse di incostituzionalità e squadrismo. Orbene, proprio chi evoca queste circostanze dimostra una scarsa frequentazione della nostra Carta fondamentale nonché preoccupanti manchevolezze della memoria. Dico, per quanti hanno tutto l'interesse a dimenticare, che il più grave fenomeno squadrista del bel Paese dal dopoguerra ai giorni nostri porta il nome di Volante Rossa, cioè quella polizia dell'allora Partito comunista italiano dotata di armi e di divise che, a differenza delle pacifiche ronde odierne, venne istituita non per prevenire reati, ma per commetterli. peso, lo dice anche un famoso regista tanto amato dalla sinistra. Occorrerebbe perciò un certo pudore nel proferirne alcune che evocano atroci scenari e per qualcuno sarebbe opportuno arrossire nel pronunciarle. Quanto alla Costituzione, ebbene, confesso di non amare la vuota retorica di chi le ruota intorno il turibolo, incensandola e venerandola come fosse un libro sacro. Il testo elaborato dai Costituenti non scaturisce da rivelazione divina e, come tutte le leggi scritte da uomini, anche la nostra Carta fondamentale è criticabile, perfettibile, opinabile. Tuttavia, in essa risiedono principi di libertà che risultano ragionevolmente indiscutibili nella loro intangibilità, come il diritto di associarsi liberamente. La Costituzione, all'articolo 18, sancisce: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale». Ebbene, forse qualcuno tra gli sputasentenze che bollano di incostituzionalità le ronde dei cittadini ritiene che al singolo individuo sia proibito incamminarsi per la propria città e segnalare eventuali reati o potenziali situazioni di pericolo alle forze dell'ordine? Sommessamente, invito quanti temono più la libertà di azione degli onesti che quella dei malfattori a riflettere anche sul fatto che il nostro ordinamento attribuisce al privato cittadino la facoltà d'arresto in flagranza di reato; questo significa che la legge riconosce al soggetto un ruolo attivo nella tutela della civile convivenza: ogni cittadino per il legislatore è in se stesso una ronda, anzi un supplente della forza pubblica qualora le contingenze lo rendano necessario. E tuttavia - lo ribadisco allo scopo di prevenire qualsiasi speculazione intorno alle mie parole ciò che la Lega Nord propone per il volontariato civico in materia di sicurezza è la semplice funzione di allertamento dei tutori dell'ordine, incombenza oltretutto attribuita precipuamente ad elementi che abbiano maturato un'esperienza specifica nel settore della pubblica sicurezza: mi pare che un ex carabiniere o un ex poliziotto possano garantire una certa affidabilità nel comporre al telefono cellulare il numero del "112" o del "113"; e lo dico con amara ironia, di fronte a tante insulse accuse, senza per altro sminuire l'importanza del compito di questi volontari. Poiché sulle ronde sono piovuti strali da ambiti ecclesiastici erranti, visto che la Santa Sede li ha repentinamente corretti, e da conventicole della sinistra, vorrei concludere queste riflessioni sul volontariato di sicurezza citando il glorioso Corpo delle pattuglie cittadine, storica ronda civica nata ed attiva a Bologna, proprio ai tempi dello Stato Pontificio e che ha continuato ad operare sino ai giorni nostri con la benedizione di vescovi e sindaci di sinistra. Per l'esattezza, vi fu un periodo in cui a tali benemeriti cittadini venne impedito di pattugliare la città: arrivò il fascismo, colleghi senatori, a sciogliere queste ronde, colpevoli di eccessiva spontaneità agli occhi del regime, un dettaglio della storia che dovrebbe ispirare profonde riflessioni. Concludo dicendo che ben vengano l'inasprimento della pena e l'effettiva espiazione, cari senatori Perduca e Poretti, così come appare opportuna l'inedita definizione di reati passionali che si sostanziano in comportamenti persecutori. Ma ogni articolato in materia di sicurezza collettiva e personale risulterà monco in assenza del completamento di norme che privilegino la sorveglianza sul territorio e il filtro agli ingressi illegali con l'adozione di strumenti efficaci, come le ronde e le vere espulsioni. Se non si chiude il circolo virtuoso repressione-prevenzione, infatti, più che la certezza del castigo apparirà rilevante la possibilità del delitto e sarà di magra consolazione vedere puniti crimini che si sarebbero potuti impedire.

la Lega preferisce prendersela con l'opposizione invece di discutere di quello che è successo nella sua maggioranza alla Camera, dove non mi risulta che noi siamo in grado di determinare alcunché. Ma questo fa comodo per non fare un'operazione verità e per non dire che all'interno della maggioranza di centrodestra ci sono opinioni legittimamente diverse.

in qualche modo ambivalente. Come sa bene il Ministro (che ringrazio per la presenza), noi siamo molto contenti che finalmente si legiferi su questo punto e che finalmente si introduca nel nostro codice il reato di *stalking*.

al Parlamento di votarlo; ma dietro di esso vi era tutto un movimento di donne, di opinione pubblica e di specialisti che richiamavano l'attenzione dei politici e dei decisori

dalle molestie persistenti e dagli atti persecutori si era già passati all'aggressione, quando non alla morte. Ricordiamo il caso eclatante di una donna uccisa dopo diversi atti persecutori trascurati dalle

Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, questo provvedimento che ci è stato trasmesso dalla Camera, ovviamente e significativamente modificato, ci porta però a discutere oggi di alcune norme residuate in materia di *stalking* e di violenza sessuale. Quindi, ci troviamo a discutere di un provvedimento comunque molto importante. Dico molto importante perché sicuramente la violenza e le molestie contro le donne sono da tempo, anche nel nostro Paese, una vera e propria emergenza. Parlo, in primo luogo, di un'emergenza sociale, testimoniata dal numero crescente di episodi di violenza registrati dalla cronaca e che spesso - e questo è uno degli aspetti più brutti del fenomeno - si consumano nel silenzio e nella segretezza dei nuclei familiari. Parliamo però anche di un'emergenza culturale, che si riflette nella diffusione allarmante di molestie e violenze nei confronti delle donne, tutto ciò in un contesto segnato purtroppo da antichi e nuovi fondamentalismi, che sempre più spesso individuano nella libertà femminile il terreno da presidiare e conquistare, anche conculcando i diritti più elementari, fino a forme di vero e proprio schiavismo delle donne e delle bambine. Non siamo dunque alle prese solo e principalmente con un problema di repressione o di ordine pubblico, ma con un'emergenza globale e, per quanto riguarda l'Italia, con un'eredità sociale e culturale che, dietro alle statistiche, rivela un ritardo grave della coscienza civile del Paese nel campo delle libertà individuali, dell'inviolabilità e della dignità del corpo femminile, della prevenzione dei reati sessuali e dell'assistenza delle vittime. In anni recenti la maggior parte dei Paesi europei ha affrontato con legislazioni specifiche il problema, in misura diversa e nel rispetto delle singole specificità, intervenendo in modo efficace

misure di contrasto, con un rafforzamento della tutela penale (ma questo in qualche modo nel provvedimento c'è), nonché misure volte ad una migliore tutela delle vittime in ambito processuale. Purtroppo questo non è avvenuto, lo abbiamo già detto: mi auguro che il Governo e il Parlamento possano ben presto ritornare sul tema e affrontarlo nel suo complesso,

violenza e soprattutto (voglio ricordarlo) all'interno di una relazione affettiva e delle mura domestiche. I dati ci dicono che ancora una volta a perpetrare la violenza è quell'uomo di cui le donne si sono fidate, che hanno amato e che dice di amarle; tuttavia, per una donna che trova il coraggio di denunciare, quante altre subiscono in silenzio vessazioni, violenza psicologica, fisica e sessuale? Sono tante, tantissime; per questo, dunque, le misure repressive non sono sufficienti. C'è un problema legato ai valori, torno a ripeterlo: la famiglia è cambiata, ma restano i valori tradizionali legati ad un modello tradizionale patriarcale, per il quale la donna si trova immersa in una violenza simbolica, che si adatta male ai cambiamenti delle relazioni tra sessi nel mondo occidentale. L'esaltazione della famiglia scoraggia le donne: chi subisce una violenza nelle mura domestiche si vergogna a uscire e a dire che la sua famiglia non funziona, perché il modello le dice che la famiglia va tutelata. Signor Ministro, concludo il mio intervento con una preghiera che rivolgo a lei, e idealmente al ministro Maroni, anche se oggi non è presente in Aula. Abbiamo detto che ci sono delle pene severe per la repressione di questo tipo di reati, che le forze dell'ordine tuteleranno le nostre donne per le strade, anche quelle che subiscono violenza tra le mura domestiche. Il ministro Maroni ha parlato più volte di un aumento del 10 per cento rispetto al 2008 delle risorse per il comparto sicurezza: peccato che pochi giorni fa gli esperti delle principali organizzazioni sindacali del settore hanno avuto modo di puntualizzare

affinché i nostri organismi di pubblica sicurezza siano dotati di strumenti e risorse adeguate, non solo a consentire loro una preparazione specifica che è necessaria in questa materia, ma anche a disporre di strumenti per intervenire efficacemente nel settore.

dobbiamo obiettivamente concordare - sono divenuti una nuova piaga per la nostra società. Recriminiamo sul fatto che la Camera abbia bocciato due norme importanti e cardine

possibilità di essere fermati fino a 180 giorni nei Centri di identificazione e di espulsione. Oggi sappiamo che dobbiamo approvare questa normativa monca, un provvedimento zoppo:

puntare i piedi su queste norme in funzione delle direttive comunitarie, l'ultima delle quali è la n. 115 del 2008, che disciplina effettivamente l'espulsione degli stranieri consentendo fino a 18 mesi la detenzione in centri di accoglienza.

cento della popolazione, è questa la quota degli stranieri, commette quasi la metà di questo tipo di reato.

Diciamo che in questa fase non possiamo non vedere il vero aspetto della situazione, cioè per il rischio di vederci appioppato il termine di xenofobi non possiamo far finta di non vedere la realtà per quella che oggi è. Che valutazione abbiamo fatto della vicenda? Qui dobbiamo scomodare Beccaria, che già due secoli fa ci lasciò in eredità degli interessanti studi: il primo sulla certezza della pena l'efficacia sta non tanto nel comminare pene altissime, ma nell'essere in grado di far scontare questo tipo di pena. Beccaria, però, ci ha lasciato altri tracciati. Ricordo "Dei delitti e delle pene", concernente la funzione della pena,

del nostro sistema, cioè la certezza della pena che - ahimè - oggi non c'è più. Qual è la novità introdotta? Diciamo che per certi reati, giudicati gravi e di gravissimo allarme sociale, gli sconti giudiziari non si applicano. È chiarissimo! Così, di fatto, si persegue proprio l'obiettivo che si diceva: efficacia della norma, efficacia della sanzione, certezza della pena e il cerchio chiude! In sostanza, per reati di violenza sessuale, atti sessuali su minori, violenza sessuale di gruppo, oltre a tutti quelli rientranti nell'articolo 51, (mantenimento in schiavitù, pornografia minorile, traffico di sostanze stupefacenti), la regola sarà la custodia cautelare in carcere. Nessun tipo di beneficio!

entro 60 giorni dallo sbarco, cioè non ancora identificati per mancanza di tempo perché si è cassata quella famosa norma prevista dei 180 giorni per il trattenimento nei centri di espulsione ed identificazione? Qui parliamo, colleghi, non colleghi, non di ideologia politica ma di un bene comune, cioè la sicurezza di tutti i cittadini, soprattutto in questi casi dei più deboli (minori, donne e disabili). Pertanto, noi esortiamo innanzitutto ad approvare questa legge perché è impellente, ma quanto prima dovremo anche ripristinare quelle norme inopportunamente e sciaguratamente cassate, che servono al nostro sistema. Grazie

al contenuto di questo intervento, di non toccare il tema dell'automatismo cautelare contenuto nella norma che estende ai reati di natura sessuale l'obbligo di custodia cautelare in carcere. Mi vedo quasi costretto a fare un'annotazione su questo punto, avendo, qualche istante fa, sentito parlare di certezza della pena come base concettuale di questa norma. Allora, si può discutere di tutto col massimo rispetto dei punti di vista diversi, ma bisogna avere la massima chiarezza sui concetti: la certezza della pena con la custodia cautelare non c'entra nulla. *(Applausi dal Gruppo PD).* La certezza della pena riguarda la pena successiva ad una sentenza passata in giudicato; la custodia cautelare in carcere, obbligatoria o meno, riguarda un procedimento in corso, normalmente nella fase delle indagini preliminari. Poi possiamo discutere del fatto e dell'opportunità di istituire un meccanismo che, dal punto di vista della ingegneria processual-penalistica, è da tutti considerato assai rozzo e che spesso produce gli effetti opposti; ma non è il mio intento in questo momento. In questo intervento di breve durata, che cerca di toccare alcuni dei temi importanti del decreto‑legge al nostro esame, il mio intento è quello di dire: cerchiamo di intenderci sulle cose di cui parliamo: con la custodia cautelare la certezza della pena non c'entra nulla. Detto questo, vorrei fare alcune brevi notazioni, non prima di aver espresso soddisfazione per il fatto che, comunque sia, secondo una procedura che non ci entusiasma ed un itinerario parlamentare che poteva essere più lineare, siamo oggi qui a parlare di un'innovazione normativa importantissima e veramente urgente; tanto urgente che abbiamo tentato di introdurla in precedenti provvedimenti che avevano a che fare con la sicurezza collettiva e ci è stato risposto, per l'appunto, che si trattava di materia che sarebbe stata elaborata e trattata in un disegno di legge.

politica generale in materia di sicurezza e di gestione delle risorse giudiziarie di polizia da parte del Governo e della maggioranza. C'è una norma, quella di cui all'articolo 6, in cui si affrontano parecchie questioni; fra queste è toccato il tema importante della videosorveglianza nei luoghi pubblici.

c'è un però - contemporaneamente alla redazione di questo decreto-legge ed alla sua proposizione nella sede parlamentare, il Governo ha elaborato e proposto un disegno di legge in materia di intercettazioni nel quale vi sono molte amenità - non è questa la sede per parlarne - e, fra queste, la previsione di una complessa procedura giudiziaria per autorizzare le riprese anche in luoghi pubblici da parte della polizia giudiziaria.

colleghi leghisti, ad un meccanismo potente di controllo del territorio con le videoregistrazioni, ma l'impossibilità di utilizzarle perché la normativa sulle intercettazioni telefoniche, ambientali e visive che vi apprestate ad approvare - o che renderebbe, per difetto di quella complessa e farraginosa procedura giudiziaria, inutilizzabili tali riprese. È bene chiarirsi le idee, è bene aver chiaro chiaro che questi temi si affrontano con una strategia, non decidendo ogni mattina che norma buttar giù, per esigenze, a volte - duole dirlo - di propaganda politico-elettorale. La norma chiave di questo testo normativo è quella che prevede il reato di *stalking*, cioè di persecuzione assillante. Siamo contenti che ci sia, un po' meno di com'è concepita: essa presenta diversi aspetti aspetti difettosi dal punto di vista della tecnica legislativa e diversi profili di mancata conformità al precetto penalistico della determinatezza della fattispecie, in particolare laddove si prevede che il reato sussista quando la condotta genera un perdurante e grave stato d'ansia o di paura; trattasi di condotta descritta in maniera imprecisa, che richiederebbe, o richiederà, una serie di accertamenti, spesso complessi, a volte impossibili, e che noi suggeriamo di cambiare con un emendamento di cui discuteremo al momento opportuno. problemi con la perseguibilità a querela, che in un caso come questo è conveniente ma che deve avere il temperamento dell'irretrattabilità (ed anche in questo caso proponiamo un emendamento di cui discuteremo). problemi con l'individuazione dei soggetti che possono porre in essere questo tipo di condotta, in particolare laddove è escluso che essa sia posta in essere dai soggetti che statisticamente più spesso

Signora Presidente, signora Ministro, colleghe e colleghi, il retaggio culturale della donna oggetto nella società odierna, almeno in quella occidentale, lo sentiamo superato o almeno è questo il nostro sentimento. La La strada per giungere a questo risultato, ma che nei fatti considero quasi un diritto, non è stata certamente facile. Ci sono volute tante battaglie e molte donne coraggiose. Per questo, permettetemi di fare gli auguri ad una donna che

Il testo oggi alla nostra attenzione ci offre dunque la grande opportunità di continuare sul percorso dell'affermazione di un importante diritto per la donna: quello di non essere considerata al pari di un oggetto.

La straordinaria valenza culturale di questo provvedimento normativo la si apprezza ancora di più alla luce degli efferati episodi degli ultimi mesi nei confronti di donne e ragazze poco più che bambine. Introdurre nel nostro ordinamento misure per assicurare una maggiore tutela al bisogno di sicurezza della collettività, ed in particolare a fronte dell'allarmante crescita di episodi collegati alla violenza sessuale, è un risultato straordinario che tutte le colleghe ed i colleghi spero vogliano condividere. Lo si vuole anche ritenere un primo ma fondamentale passo verso una più ampia legge sulla quale il Parlamento lavora e continuerà a lavorare. Grande è, dunque, l'importanza di questo testo, che prevede un sistema coordinato di norme finalizzate al contrasto di questi fenomeni ed una più concreta tutela delle vittime. Inoltre, riprendendo il testo approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati il 29 gennaio scorso, si prevede anche l'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori. La violenza fisica e sessuale rappresenta la più bieca violazione dei diritti umani, talmente grave da aver suscitato l'attenzione dei Governi e da farla emergere come una delle priorità. Nelle nostre società moderne e democratiche, in cui i diritti delle donne dovrebbero appartenere a quel patrimonio di diritti universali, dobbiamo rilevare il dato sconfortante della violenza come una tra le prime cause di morte nel mondo per le donne tra i 16 e i 44 anni. In Italia dati dell'ISTAT hanno la portata di un vero bollettino di guerra. Oltre 6 milioni sono le donne vittime di violenza fisica, 5 milioni di queste hanno subito violenze sessuali, 1 milione le donne che hanno subito stupri o tentativi di stupro, 2 milioni le donne che hanno subito comportamenti persecutori, comunemente conosciuti come *stalking*. Purtroppo nell'odierna società in cui è diventata dominante la dittatura dei desideri, è assurto a divertimento stuprare una giovane ragazza appena conosciuta, anche solo per passatempo, così come diventa normale aggredire una giovane coppia chiudendo nel bagagliaio l'uomo e violentando la giovane compagna. Spesso non c'è neppure la giustificazione della degradazione morale e materiale in cui vivono le persone che si macchiano di questi reati per spiegare tali soprusi; spesso si tratta solo di ricerca di trasgressione, di emozioni forti, del desiderio di sopraffare, di umiliare, di voler imporre la legge del più forte sul più debole. violenze di gruppo, gli atti di bullismo sono frutto di una mal posta concezione di libertà scambiata per licenza, sciupando le cose belle della giovinezza, violando, con forza vile e spesso impunita, il corpo e lo spirito delle proprie coetanee. Viviamo questo paradosso: da un lato sosteniamo con tante azioni positive la cultura dei diritti umani, mentre dall'altro si pratica una non cultura, quella che afferma una visione della sessualità come sopraffazione, desiderosa solo di prendere quello di cui si ha voglia. Ecco perché nel presente decreto tanta attenzione viene posta all'educazione, all'aspetto culturale, soprattutto a partire dalle scuole per tentare con pazienza, ma anche con grande determinazione, di riannodare il filo strappato della cultura del rispetto dell'altro. Forse è anche arrivato il momento in cui siamo chiamati ad un serio esame di coscienza, in questa società così liquida, dove regna l'estraneità, dove non esistono più i rapporti di vicinato, in cui è più facile non ascoltare ciò che avviene nella casa accanto o accettare per buona la scusa di una banale caduta per giustificare un vistoso ematoma ricorrente. Eppure, sappiamo che esiste una vera e propria emergenza silenziosa che vede le donne oggetto di abusi soprattutto all'interno delle mura domestiche. di esse non denuncia la violenza perché spesso vive in una condizione di solitudine familiare e di relazioni e non sa come poterne uscire; spesso subentra un senso di vergogna, di colpa, si arriva persino a pensare di essersela cercata e voluta. Questa violenza dal volto amico è la più dolorosa e destrutturante. Così come inquietante è il reato di *stalking*, il piacere di perseguitare e infliggere sofferenza, il voler dimostrare di sentirsi più forti e padroni di riprendere il proprio spazio nella vita della persona che ha scelto invece di troncare o non accettare un rapporto. Erano anni che si parlava di *stalking* e finalmente anche in Italia si sono prese misure per contrastare questo fenomeno che in altri Paesi, quali ad esempio gli Stati Uniti, è riconosciuto come reato già da 15 anni.

È importante, dunque, che vi siano leggi che rafforzino nel nostro Paese la percezione di legalità da parte dei cittadini che si aspettano una legge chiara che non lasci spazio ad interpretazioni e quindi a possibili impunità per i trasgressori, una legge efficace, non ambigua, non soggetta a trattamenti arbitrari in fase di applicazione, una legge capace di garantire e tutelare gli onesti, gli indifesi, i deboli e le donne. donne. La legge ha sempre anche una valenza educativa e in questo senso resta l'unico strumento potente. Oggi con ragione possiamo ritenerci soddisfatti e attraverso il nostro voto cercheremo di cambiare quella parte oscura che ancora è presente nella nostra cultura, quella parte della società che disprezza la mitezza, la solidarietà, il rispetto dell'altro, la sobrietà dei comportamenti.

Presidente, interverrò brevemente prendendo atto della soddisfazione complessiva manifestata dall'Aula su una tematica di particolare importanza e dando atto che la tematica era stata affrontata anche nella scorsa legislatura. bisogna considerare che un conto è dire, discutere, presentare disegni di legge, altra cosa è intervenire con urgenza con un decreto-legge rendendosi conto che, nel vuoto normativo, gli abusi e gli attacchi nei confronti delle donne in particolare, erano diventati talmente insopportabili da far sì che un Governo che guardi veramente con attenzione particolare a tutte le problematiche intervenisse con un decreto-legge, quindi, con norma immediatamente applicabile applicabile dalla magistratura. È evidente che qualsiasi norma è perfettibile. Anche in questa occasione, se si fosse rispettato l'equilibrio dei tempi tra Camera dei deputati e Senato, sicuramente sarebbero state evitate tante discrasie. Probabilmente lo stesso reato previsto dall'articolo 612-*bis* si sarebbe potuto confezionare in modo anche più incisivo, in modo più applicabile, in modo più forte, a tutela delle donne e a tutela di tutti. è altrettanto vero che vi sono altri disegni di legge in discussione alla Camera ed al Senato in cui, comunque, dopo una prima messa alla prova, dopo una prima possibilità di test, si possono

una maggiore certezza della pena nel momento in cui si riferisce, mediante l'articolo 3, al venire meno di alcuni benefici penitenziari e, quindi, della possibilità di

il problema della videosorveglianza. Posso però precisare fin da ora che mentre nel disegno di legge sulle intercettazioni la ripresa video è mirata

Il problema dell'investimento nelle risorse per la prevenzione probabilmente è anche più importante di quello della repressione, perché quando si arriva alla repressione il danno è già stato compiuto.

crea un problema non solo di sovraffollamento ma di concreta attuazione dell'attività amministrativa di identificazione, anche eventualmente ai fini di un asilo politico.

facile pensare che essi possano essere preda di coloro che sfruttano i lavoratori tramite il cosiddetto lavoro nero, se non anche della criminalità organizzata. Comunque costoro qualcosa dovranno fare per poter mangiare ogni giorno.

Non vi è alcuna norma di legge che vieti ad un gruppo di cittadini italiani, in qualsiasi ora, in qualsiasi strada, in qualsiasi città della Repubblica italiana, di andare in giro per verificare se succede qualcosa e, con senso civico, avvertire le forze dell'ordine o le ASL o eventuali organismi pubblici. Quindi, non vi è assolutamente alcuna necessità di questa polemica perché non si è parlato di nessuna

Vi sono degli esempi illustri. Ne hanno citato i colleghi: parliamo dei Barracelli, dei *City Angels*, delle pattuglie cittadine di Bologna, ma anche delle ronde dei commercianti che in Sicilia, a Capo d'Orlando e a Palazzolo Acreide, insieme alle forze dell'ordine hanno sconfitto il *racket* delle estorsioni. Ipotizzare e anche prevedere normativamente una partecipazione attiva dei cittadini alla problematica dell'ordine pubblico e non uno scarica barile esclusivamente sulle forze dell'ordine e sulla magistratura, potrebbe probabilmente essere un buon esempio di educazione civica e di partecipazione attiva alla migliore gestione della legalità e della sicurezza.

fornito spunti di riflessione utili alla discussione generale, al dibattito e alla valutazione complessiva di questo provvedimento. vorrei ribadire la necessità di intervenire con un decreto‑legge perché credo che lo Stato avesse il dovere di dimostrare con fermezza e senza equivoci di essere a fianco di quelle donne che non hanno avuto alcuno strumento, o ne hanno avuti di insufficienti, per potersi difendere contro quegli atti efferati ed odiosi che costituivano una minaccia per la vita di tante, di troppe donne nel nostro Paese. È vero che c'è stata fortunatamente una diminuzione dei casi di violenza sessuale, ma questo non vuole dire che ci sia stata una diminuzione dell'efferatezza e dell'odiosità di questi atti che il Governo ha deciso fin dal suo insediamento di contrastare con grande determinazione e con grande efficacia. dai numeri: gli arresti per*stalking* da quando il decreto‑legge è entrato in vigore sono arrivati a 102 e sono 132 le persone denunciate,

Ho ascoltato attentamente gli interventi dei colleghi senatori e riguardo alla necessità di un'azione più generale riguardo alla necessità di un'azione più generale di informazione, di sensibilizzazione, di rafforzamento della tutela penale sono in grado di rassicurare i colleghi, perché

le pubblicità che riguardano il numero verde antiviolenza "1522", che presto diventerà numero verde anti*-stalking*. Ebbene, dall'entrata in vigore del decreto‑legge, le telefonate sono aumentate per cento, segno che le donne hanno capito che possono denunciare perché finalmente trovano tutela da parte dello Stato. Sono poi anche da ricordare le azioni del Dipartimento per le pari opportunità che mirano a finanziare l'attività dei tanti centri antiviolenza che sono presenti sul territorio. Lo stesso decreto‑legge che ci apprestiamo ad approvare prevede un incremento del fondo antiviolenza fondo antiviolenza di 3 milioni di euro, che verranno impiegati proprio per azioni di prevenzione di questi atti particolarmente odiosi e di tutela delle vittime di atti persecutori e di violenza sessuale. senatore Centaro ha poi illustrato egregiamente i tanti punti del decreto che, insieme all'introduzione del del reato di atti persecutori, costituiscono, come più volte abbiamo detto, una mano tesa verso quelle donne che subiscono quotidianamente atti di violenza anche psicologica all'interno delle mura domestiche. Tante sono le misure che possono e devono essere considerate a tutela e a favore delle donne che subiscono violenza: l'obbligo di custodia cautelare in carcere; la limitazione dei benefici premiali; l'arresto obbligatorio in flagranza con la possibilità poi di procedere con il rito per direttissima; il gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale, sia una misura di equità e giustizia, ma anche che aiuterà le tante donne che per mancanza di mezzi economici non denunciano ad uscire della solitudine e, soprattutto, dal silenzio e a denunciare gli atti di violenza cui purtroppo quotidianamente devono sottostare.

alle donne dignità, sicurezza e libertà, perché credo che sia inutile parlare di pari opportunità nel mondo del lavoro e in politica se prima di tutto non ci preoccupiamo di assicurare alle donne quella sicurezza e quella dignità che quotidianamente vengono messe in discussione da atti che sono da condannare con grande fermezza e decisione. Il Governo l'ha fatto e lo sta facendo perché ha posto come priorità della sua agenda politica la lotta contro la violenza sessuale e contro ogni forma forma di violenza. Credo che la lotta alla violenza sessuale o si predica o si fa: questo Governo ha dimostrato di volerla fare e la sta facendo.

«La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

parere non ostativo nel presupposto che alla disposizione di cui all'articolo 4 si proceda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12-*ter*.0.4 e 6.1. In ordine alle proposte 11.0.4 e 12-*ter*.0.6, il parere è non ostativo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che al comma 1 la parola: "istituiscono" sia sostituita, con le seguenti: "possono istituire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente";

«In ordine alla proposta 11.0.1, il parere è non ostativo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che dopo la parola: "programmano" siano inserite le seguenti: "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente". In ordine alle proposte 12-*ter*.0.2 e 12-*ter*.0.3, il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. In ordine alla proposta 12-*ter*.0.7, il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che al comma 1 la parola: "istituiscono" sia sostituita dalle seguenti: "possono istituire". Il parere è di semplice contrarietà in ordine alla proposta 11.0.7. In ordine agli emendamenti 4.1 e 4.2, il parere è non ostativo nel presupposto, in relazione a quanto osservato sul testo, che si proceda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Il parere è infine non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

non armati» dovrebbe recitare: «al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale».

del 2009 sono state soppresse le richiamate disposizioni dell'articolo 6, commi 3-6», in quanto non ci fu un voto; il dispositivo dovrebbe essere così modificato: «in sede di approvazione, alla Camera dei deputati, dell'AC 2180, a confermare le disposizioni sull'utilizzo delle forme di volontariato finalizzate allo svolgimento di attività di osservazione del territorio ai fini della segnalazione agli organi di polizia locale, ovvero alle forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale con una presenza sul territorio aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalle forze dell'ordine e di polizia statali e locali.

all'ergastolo e quindi vorremmo eliminarlo dal decreto sulla sicurezza. In seconda battuta, se proprio si ritiene l'ergastolo assolutamente necessario, vorremmo che i crimini in questione fossero esplicitamente collegati.

la possibilità che venga introdotto e previsto l'ergastolo per questo tipo di reati. L'emendamento cerca di

È una correzione di tipo apparentemente lessicale, ma che prevede invece una contestualità cronologica e, quindi, la necessità di cambiare la formulazione. Più in generale, sono emendamenti che cercano di evitare la pena dell'ergastolo, in coincidenza in concordia con quanto prevede la nostra Costituzione. Di conseguenza, le pene dovrebbero tendere alla rieducazione del condannato. Per di più, lo scorso novembre il Commissario europeo per i diritti umani ha precisato come sia necessario un riesame in merito al ricorso all'ergastolo. Il Commissario europeo per i diritti umani ha infatti criticato l'esistenza dell'ergastolo e questa critica diventa tanto più forte, dal dal punto di vista dei cittadini dell'Unione europea, sulla base dell'integrazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del Trattato firmato a Lisbona. Noi, invece, andiamo nella direzione esattamente opposta e prevediamo nuove fattispecie per cui è previsto

leggermente superficiale e generale sulla certezza della pena, ma non è questa la questione in discussione. La pena viene comminata a seguito di un processo,

2, comma 1, lettera *a)*, sarebbe quanto mai doveroso prevedere una significativa contrazione dei tempi massimi di custodia cautelare per quasi tutte le ipotesi di reato previste, al fine di non sacrificare per periodi eccessivamente lunghi la libertà personale del cittadino imputato, che in quanto tale è presunto innocente fino alla sentenza definitiva.

chiediamo la soppressione dell'articolo 3, perché l'esclusione dei benefici penitenziari, presupponendo una presunta pericolosità sociale individuata solo in base al titolo di reato, ossia in virtù di un tipo di autore, si pone in evidente contrasto con i princìpi cardine del nostro sistema costituzionale, tra i quali si iscrive certamente la finalità rieducativa della pena. Peraltro, tale deroga ai principi contenuti nella legge Gozzini, indiscutibile baluardo dei diritti civili dei detenuti, sembra preludere ad altri futuri possibili interventi di modifica della legge stessa, con il rischio di vanificare l'indubbia e proficua capacità di risocializzazione dimostrata dalle misure alternative al carcere.

è il ricorso a strumenti del tutto inadeguati, destinati a cadere, a nostro giudizio, sotto il vaglio di una verifica di costituzionalità. È un aspetto molto delicato: in queste norme si afferma che non potranno essere concessi benefici se non a condizione che vi sia una collaborazione giudiziaria, collaborazione che richiama che richiama l'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. Questo è un uso scorretto, errato e dannoso di istituti che vengono concepiti per ben altre finalità, quando si può ricorrere invece a strumenti - come quelli che noi proponiamo - che siano più adeguati allo scopo da raggiungere. L'articolo 4-*bis* della legge n. legge n. 354 del 1975 è stato introdotto, insieme all'articolo 41-*bis,* per contrastare il crimine organizzato, la cui natura, capacità di penetrazione e offensività verso i beni tutelati dalla legge sono ben noti.

spazzate via dal nostro ordinamento giuridico dalla Corte costituzionale è per la necessità di contrastare il crimine organizzato.

che la concessione di benefici carcerari sia subordinata innanzitutto all'organizzazione e all'espletamento di procedure e programmi che tendano al recupero del detenuto: non parliamo di metodi barbarici di metodi barbarici o di castrazione, ma di recupero anche del reo di questi odiosi delitti attraverso procedure che devono essere realizzate da organismi competenti. A seguito dello sviluppo e dell'attuazione di queste procedure, si dovrà vagliare in maniera seria e adeguata se il soggetto

riteniamo che questa sia una norma elettoralistica, che sfiora la demogagia ed il populismo: concedere a chiunque il gratuito patrocinio indipendentemente dal reddito francamente è è inspiegabile anche perché andrebbe a mettere le condizioni di una concessione automatica dello stesso. Forse sarebbe stato più ragionevole prendere in considerazione la cifra, che

soltanto in parte, ciò che dice il senatore Perduca, vorrei ricordare che abbiamo dato parere favorevole alla norma sul gratuito patrocinio per le vittime di stupro quando ci siamo pronunciati sull'Atto Senato n. 733 poco tempo fa. fa. A questo punto ripercorro la stessa argomentazione: poiché gli stupri avvengono anche in ambito familiare e noi stiamo parlando qui di reati che toccano la violenza domestica, oltre che lo stupro e lo *stalking*, e che sono tutti imparentati tra loro, l'estensione del gratuito patrocinio a tutte le vittime ed in particolare alle donne è un segnale di attenzione nei confronti delle vittime da parte dello Stato.

avessimo previsto un'aggravante per gli apparentati. Ma qui si prevede l'aggravante soltanto per i non apparentati. Quindi, la motivazione, per quanto comprensibile e - ripeto - generalmente condivisibile, avrebbe dovuto trovare

Presidente, ricordo al senatore Lusi che l'ottimo è nemico del bene, che il decreto scade il giorno 25 aprile e che comunque una modifica può essere sempre realizzata successivamente; questo peraltro dà conto del disequilibrio dei tempi di trattazione tra Camera e Senato. LUSI

Senatrice Incostante, mi scusi, questo vuol dire che lei trasforma l'emendamento in un ordine del giorno?

sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. Il discorso è analogo perché si fa riferimento all'autorizzazione agli enti locali ad utilizzare in luoghi pubblici o aperti al pubblico sistemi di videosorveglianza. La norma, così come è formulata, desta qualche perplessità, sia per quanto concerne i principi di riserva di legge e di tassatività, ma anche in relazione alle modalità.

si chiede se questi dati saranno acquisiti secondo le norme relative ai tabulati telefonici oppure ai sensi dell'articolo 234 del codice di rito e dunque in quanto semplici documenti.

in materia di videosorveglianza e conservazione dei dati impongono una serie di requisiti per la legittimità delle relative operazioni. Quindi, tali norme e requisiti dovrebbero comunque essere richiamati anche perché

con l'orientamento espresso ripetutamente dalla Corte di cassazione e da ultimo dalle sezioni unite nel 2006. Ciò dà dunque l'idea di un Governo legislatore che in questa materia ha dovuto quasi tappare i buchi e navigare al buio

G6.102 affronta il tema delle risorse destinate al comparto sicurezza.

nuovamente con norma cosiddetta interpretativa eliminando dalle somme che possono essere distribuite i proventi della gestioni dei beni e delle aziende confiscate, ossia si riducono ulteriormente

si prevede che nei prossimi anni, nel prossimo biennio, a causa del *turnover* altre 12.000 unità verranno a mancare perché andranno in pensione. Al riguardo il Governo non ha predisposto strategie di intervento,

questa si riferisce alla videosorveglianza di un territorio, di luoghi aperti pubblici, di luoghi pubblici eccetera, quella si riferisce all'invasione della *privacy* di un determinato soggetto che viene ripreso in quel momento. Dunque vi è una differenziazione di carattere soggettivo e oggettivo. Per quanto attiene poi alle indicazioni del collega Li Gotti, preciso che con questo decreto-legge vengono stanziati 100 milioni di euro alle necessità delle forze dell'ordine, sono, ad esempio, previste assunzioni di ufficiali da parte dell'Arma dei carabinieri, quindi vi è un intervento chiaro e preciso nel senso della sicurezza e del controllo del territorio.

invece, si fa riferimento alla videosorveglianza e alla disciplina conseguente, cui ha fatto riferimento il senatore Mazzatorta, sotto il profilo della conservazione.

in data 9 aprile 2009 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, ha approvato un decreto che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 2.875 unità 2.875 unità di personale nelle forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco. Per tale ragione il parere sull'ordine

Ciò che determina la crisi del sistema sicurezza non è la sicurezza sussidiaria o complementare, né sono i protocolli che i sindaci possono promuovere con i rondisti di varia natura che servono solo a caricare di un ulteriore onere finanziario gli enti locali i quali, comunque, dovranno sostenere almeno il costo del rimborso delle spese di questi cosiddetti volontari della sicurezza urbana. modo il cittadino sarà chiamato a pagare due volte per lo stesso servizio: una volta allo Stato, che per Costituzione deve occuparsi dei compiti relativi alla sicurezza, e una volta ai sindaci, ai quali, per esercitare i poteri che esercitano, non avendo i vigili urbani e non prevedendo

con i carabinieri in pensione o con qualche associazione per risolvere la questione. Questo tema fortunatamente è scomparso dal decreto. Ci saremmo augurati che, al di là del reclutamento per tre anni di un certo numero di unità presso l'Arma dei carabinieri, fosse stato previsto un finanziamento consistente delle forze

invertire la tendenza in forza della quale non è possibile costruire un sistema della sicurezza fatto solo ed esclusivamente di annunci e di militari che passeggiano, anche perché i militari costano più

allora ero alla Camera, però la stessa cosa era avvenuta al Senato - un emendamento analogo che comprendeva più o meno queste cifre e presupponeva la possibilità di assumere, laddove esistevano molte deficienze d'organico,

per quanto riguarda le somme confiscate che si vogliono destinare per 200 milioni, che non esistono nemmeno i 100 milioni, che solo alla fine del 2009 forse saranno presenti nelle casse. Tant'è vero che in Commissione giustizia alla Camera era stato approvato l'emendamento Vietti che portava a 150 milioni, ma poi è stato proposto l'emendamento dal Ministero dell'economia perché in cassa non c'erano i soldi per poter sostenere quella proposta. Quindi, nel fondo giustizia, tra le somme confiscate non esistono queste cifre; per cui correttamente la Commissione bilancio ha dato parere contrario.

Presidente, poiché alla Camera si sta discutendo la nuova disciplina sulle intercettazioni, che che riguarda anche la disciplina delle riprese televisive e quanto altro, credo che il tema dell'ampliamento dei sistemi di videosorveglianza di cui possono avvalersi sindaci ed enti locali locali dovrebbe essere stralciato da questa materia e inserito nell'ambito della discussione che più propriamente e generalmente si sta facendo sulla questione, almeno per due ordini di ragioni. della rilevanza probatoria delle videoriprese fatte dai Comuni. La disciplina che noi abbiamo in questo testo non chiarisce qual è il rilievo probatorio di queste riprese.

alla Camera. Dunque, ritengo sarebbe più opportuno stralciare i commi 7 e 8 e affrontare anche il tema dell'ampliamento dell'uso dei dispositivi di videosorveglianza da parte degli enti locali nell'ambito della disciplina delle intercettazioni. Questo è il senso

Personalmente sono soddisfatta che venga approvata la normativa sullo *stalking*. Lo dico non soltanto perché ho collaborato alla scrittura del precedente testo di legge, che poi nella precedente legislatura aveva dato vita anche ad un atto condiviso,

perché probabilmente avremmo potuto già da allora dar vita ad un testo condiviso. Ora si tratta soltanto di mettere in luce questo non per una ragione di narcisismo, ma perché purtroppo sono derivate delle conseguenze

Purtroppo, è stato così e mi permetto di ribadirlo perché credo sia necessario per un senso di chiarezza e per comprendere la ragione per cui più volte siamo intervenuti, non certo per arrestare il corso di una legge che ritenevamo necessaria, perché quella legge fosse più perfetta possibile e potesse essere applicata chiaramente da parte di chi, come gli investigatori e i magistrati, cerca di tutelare le vittime e perseguire i colpevoli.

erano stati respinti gli emendamenti in materia, Barbara Brandolini, 27 anni, viene trovata soffocata dal suo ex fidanzato a Bergamo;

Naturalmente tutto questo all'esito di lunghi atti persecutori che all'epoca non costituivano reato; 19 agosto (questo è un omicidio che avviene in casa straniera, anche se in Italia), con un colpo alla testa una donna di 21 anni, Svetlana Sulejmanovic ed il fratello. La ragazza era incinta del terzo figlio e viene uccisa dal nonno secondo cui i nipoti gli mancavano di rispetto.

22 agosto, ad Arezzo, Luca Ferri, di 26 anni, strangola con una cintura la fidanzata e convivente Silvia Zanchi, che probabilmente voleva lasciarlo; a

29 agosto, a Pesaro, avviene un altro omicidio per la progressione del diritto di *stalking*; dopo il delitto l'uomo, che uccide a martellate alla testa la moglie, tenta Altri omicidi sono avvenuti, sempre per effetto di *stalking*, secondo questa ricerca che ritengo attendibile, il 2 settembre a Ravenna, l'11 settembre a Pisa, il 17 settembre a Bergamo, il 18 settembre in Calabria, il 19 settembre a Napoli, il 1° ottobre a Foligno, il 2 ottobre a Trapani, a Giano dell'Umbria il 6 ottobre, a Bovalino (Reggio Calabria) il 7 ottobre, il 9 ottobre a Roma,

serio. Credo che quando ci avviciniamo ad un fenomeno così serio come lo *stalking* abbiamo il dovere di pretendere che venga colmata una lacuna legislativa, che potevamo già colmare a luglio, ma che questo avvenga producendo un testo di legge tecnicamente corretto. Questo non tanto perché nella fase delle indagini preliminari, quando si lavora con gli indizi, non avremo la possibilità di intervenire immagino che la polizia, che mai è stata così solerte, pur avendo a disposizione il testo unico di pubblica sicurezza che le consentiva di convocare qualsiasi soggetto violento e autore dei reati, ma piuttosto perché nella fase del dibattimento e delle prove dovremo confrontarci con la possibilità di provare l'esistenza del reato, quindi effettivamente con una pena che sia certa e che deve essere applicabile. Questo è l'unico motivo per cui, rispetto al testo sullo *stalking*, abbiamo presentato degli emendamenti che cercano di migliorare il testo. Il primo punto è costituito dal fatto che, per anticipare la soglia dell'intervento penale rispetto a condotte che sono prodromiche potenzialmente ad atti più gravi, la norma finisce con l'incriminare comportamenti che scontano una certa indeterminatezza. Tutto questo potrebbe non rispondere ai canoni dell'articolo 25 della Costituzione e condurre inesorabilmente all'assoluzione. Naturalmente, è legittimo chiedersi se il giudice può ritenere che la condotta contestata abbia cagionato un perdurante e grave stato d'ansia o di paura alla vittima possa accertare delle condizioni soggettive senza nemmeno aver disposto una perizia; oppure basterà un prolungato stato di turbamento della vittima? Questo è il primo punto. Il secondo punto che mi affligge è quello della procedibilità a querela. Per il reato di *stalking* si prevede la querela salvo i casi di connessione con delitti per i quali si deve procedere d'ufficio, oppure per le ipotesi in cui la vittima sia un minore o un disabile. Naturalmente vi è un problema di coerenza sistematica, perché la previsione della procedibilità a querela del reato...

Possiamo dire che la procedibilità a querela non è accompagnata dal caso dell'irrevocabilità della querela per una fattispecie che consente l'adozione di misure coercitive. tutto questo desta perplessità, perché il giudice potrebbe aver arrestato una persona ed emesso una misura cautelare e in seguito, per la ritrattazione della querela, si verrebbe a creare una situazione estremamente difficile per chi ‑ magari ‑ ha perso anche la libertà. Questo è il secondo punto. Gli altri punti li affronterò nella giornata di domani.

Mi fa piacere intervenire dopo la senatrice Della Monica, che ha già evidenziato uno dei punti chiave di questa nuova figura di reato: gli atti persecutori, più mediaticamente conosciuti come *stalking*, che decidiamo di inserire nel nostro codice penale. Il nostro emendamento interviene nel primo e nel secondo comma. il primo comma e lo riformuliamo perché sia rispondente a quel principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale. Infatti, laddove si prevede di cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, si configura una determinazione molto vaga che potrebbe poi produrre difficoltà di interpretazione in sede di processo

non capisco perché l'aggravante non si preveda anche per gli attuali fidanzati e gli attuali mariti. Nell'elenco prima fatto dalla senatrice Della Monica sulle donne uccise

fossero stato ammazzate da ex fidanzati o da ex mariti. Io mi chiedo che senso abbia prevedere un codice del genere, un reato del genere e un'aggravante di questo tipo.

oso far presente ai senatori Poretti e Perduca, che si richiamano al principio di tassatività, come il loro emendamento 7.100

a non turbare le possibilità di soluzione interna, mentre l'aggravante, così com'è concepita, ha una ragion d'essere in prospettiva - è vero

che il reato di atti persecutori si rivolge a soggetti usciti dalla sfera delle relazioni domestiche della vittima, mentre per coloro che sono ancora nell'ambito delle relazioni domestiche vale l'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 11, del codice penale.

è morta, davvero vogliamo insistere a raffigurare la famiglia come un luogo idilliaco, dove tutto può essere riannodato, o non ci interessa invece puntare l'attenzione sulla vittima? Ci interessa soltanto il contesto degli ex

Signora Presidente, è un problema di coerenza. Si introduce la custodia cautelare in carcere come obbligatoria per i reati di violenza sessuale. A questo punto non si definisce qual è il caso di lieve entità, pur dicendosi che il caso è escluso. Questa è una forte incoerenza, anche perché lasciamo all'arbitrio del giudice - quello che non si vuole - stabilire in cosa consiste la lieve entità del fatto.

da cui si fa dipendere, come atto amministrativo, la procedibilità di un determinato reato. È come se dicessimo che se un mafioso viene ammonito, perché per le misure di prevenzione deve essere ammonito, e poi commette un reato, per esempio una violenza sessuale, questo diventa Dal punto di vista giuridico è assolutamente sbagliato. Da un punto di vista di fatto, poi, l'ammonimento apre a procedure amministrative di ricorso il Consiglio superiore della magistratura, forte dell'esperienza anche di vari magistrati italiani, che ha riunito per affrontare il problema delle violenze, ha fatto presente che ci può essere un'*escalation* della violenza: nel momento in cui una persona viene chiamata, se è un persecutore serio, può essere sottoposto ad una pressione psicologica tale da indurlo a farla poi scontare alla parte offesa. Questa è la ragione per cui proponiamo di sostituire l'ammonimento con un intervento del pubblico ministero o di modificare quantomeno la legge sulle misure di prevenzione.

peggio venuti al Governo, diciamola così; dovremo metterci mano abbondantemente. Siamo costretti a votare un provvedimento così come proposto, perché diversamente, come è stato ricordato dal relatore, tra quattro giorni questo decreto scade. Voi prevedete un aggravamento di pena qualora la persona sia stata ammonita. Ma sia stata ammonita quando? Se l'ammonimento risale a vent'anni prima, vale ugualmente? Se riguarda un'altra persona, vale ugualmente? Voi tutto questo non lo avete previsto. Prevedete soltanto la condizione soggettiva di una persona che abbia ricevuto un ammonimento. Quando si è trattato di prevedere l'aggravante di cui all'articolo 576 del circostanza in cui siano stati commessi atti persecutori nei confronti della medesima persona, quindi si è prevista l'aggravante con un'identità della persona offesa. Nel caso invece

sia una grossa lacuna alla quale dovremo porre rimedio. Inoltre, vi faccio presente che l'ammonimento è stato dichiarato incostituzionale sin dalla sentenza n. 11 del 1956: oggi si chiama "avviso". Non si può introdurre una norma che è stata cancellata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si chiama avviso ed è un provvedimento amministrativo, al quale non può essere collegato un aggravamento di pena e una procedibilità, nel senso che la Corte costituzionale ha ritenuto che, nel rispetto dell'articolo 13 della Costituzione, questi tipi di provvedimento o vengono adottati da un'autorità giudiziaria oppure non si può, con un atto amministrativo, determinare una rifluenza

con il tempo dovuto dalla Commissione giustizia, sarebbe stato modificato. Il Governo ha fatto veramente qualcosa di impresentabile.

desidererei sapere dalla Presidenza, o da qualche Ufficio che sappia darmi la risposta, se il concetto di delegazione del Partito radicale nel Partito Democratico sia istituzionalizzato ovvero sia un'espressione che i senatori Perduca e Poretti adoperano per ragioni di visibilità politica. Rivolgo questa richiesta per sapere quanto meno come io debba rivolgermi alla senatrice Poretti e al senatore Perduca. Di conseguenza, vorrei anche conoscere se a questa delegazione del Partito radicale nel Partito Democratico partecipi qualcun altro oltre ai suddetti senatori.

Signora Presidente, purtroppo la disturbo nuovamente perché 5.000 dipendenti pubblici delle comunità montane questo mese non prenderanno lo stipendio ed il

non risponde su come il Governo possa risolvere il problema della mancata approvazione del bilancio di previsione, che comporta di fatto l'impossibilità per le comunità montane di pagare gli stipendi alla fine del mese di aprile. dipendenti delle comunità montane delle Regioni meridionali hanno segnalato che non ricevono lo stipendio dall'inizio di gennaio. È inconcepibile che il Governo non risponda

e allora si parlerà delle reazioni violente dei lavoratori senza stipendio. Le segnalo, signora Presidente, che 250 famiglie abruzzesi non prendono lo stipendio esattamente per questo motivo.